Genova, la Liguria e, con esse, l'Italia intera sono state sconvolte dal tragico crollo del viadotto Polcevera. Quella mattina di vigilia di Ferragosto, circa 200 metri di ponte sono improvvisamente collassati, precipitando nelle acque del fiume, sbriciolandosi sulla ferrovia, sui capannoni e sulle abitazioni sottostanti: 43 vittime, bambini, donne e uomini, e 600 gli sfollati, questo è l'inaccettabile bilancio di una tragedia che poteva e doveva essere evitata. Il ponte Morandi è stato il simbolo di un'Italia dinamica proiettata verso un futuro di crescita e benessere. In pochi secondi si è invece trasformato nella dolorosa metafora di un Paese incapace di sconfiggere l'incuria, di custodire i propri beni e di garantire sicurezza ai cittadini. In quei drammatici momenti tutto il mondo ci ha osservato e ha visto una straordinaria capacità di intervenire nell'emergenza. Vigili del fuoco, Protezione civile, Forze dell'ordine, soccorritori e volontari, rischiando la vita e lavorando senza sosta, hanno restituito a tutti noi la speranza di poter ricostruire quel Paese immaginato dai nostri padri. Questa è la sfida che la politica deve raccogliere e alla quale quest'Aula, ne sono certa, non si sottrarrà. Genova non può aspettare; non può restare ferita e isolata. Le ripercussioni sociali ed economiche già devastanti sarebbero inimmaginabili se protratte un minuto in più del necessario. Servono tempestività, efficienza, sostenibilità e visione. Serve che il Paese sia unito. Solo così la ricostruzione del ponte potrà essere l'occasione per dimostrare che gli errori non si ripeteranno. Lo dobbiamo, prima di ogni altra cosa, alle 43 vite spezzate, in memoria delle quali vi invito a un minuto di raccoglimento.

di commemorazione. Senatori colleghi, il 24 agosto scorso ci ha improvvisamente lasciati l'*ex* senatore Emiddio Novi, giornalista e parlamentare di lungo corso. Novi è stato apprezzato come esponente della cultura meridionalista. Sia come professionista che come rappresentante dei cittadini ha saputo porre al centro dell'attenzione nazionale le problematiche sociali, economiche ed ambientali della sua terra. A lui si devono alcune tra le prime inchieste giornalistiche sullo smaltimento clandestino dei rifiuti tossici, tematica che poi affrontò con rigore anche in qualità di Presidente della Commissione ambiente del Senato. Senatore battagliero, ma sempre rispettoso delle idee e delle posizioni degli avversari politici, Novi ha saputo lasciare un segno nelle istituzioni grazie soprattutto a una peculiare predisposizione all'approfondimento, allo studio e alla divulgazione. Consentitemi anche un breve ricordo personale. Ho condiviso con Emiddio Novi tanti anni di attività parlamentare, tanti momenti. Ne ricordo con affetto l'equilibrio, la passione civile, l'impegno quotidiano al servizio del Paese. Mi ha sempre stupito la sua capacità di intervenire in quest'Aula con determinazione, preservando allo stesso tempo una riconosciuta oggettività di valutazione. Il suo naturale e radicato garantismo rappresenta, forse meglio di ogni altra considerazione, la sua cifra politica. Alla moglie Pina, ai figli Enrico, Alessandro e Vittorio, alla sorella Maria, che sono presenti oggi in tribuna, esprimo il mio sincero cordoglio e quello dell'intera

intervengo sulla scomparsa improvvisa di Emiddio Novi, nella certezza di interpretare e di poter condividere con tutti voi il senso di un cordoglio davvero profondo. Come molti di voi, ho avuto il piacere, anzi il privilegio, di conoscerlo e di frequentarlo. Ho avuto la possibilità di condividere con lui anni e anni di battaglie politiche comuni, ho avuto modo di apprezzarne la straordinaria intelligenza, la profonda cultura, la sua particolare perspicacia politica, il suo alto senso dello Stato, la sua costante volontà di servire e battersi per il Paese, ma soprattutto per i più poveri e per i più deboli, la sua capacità di saper sempre offrire al dibattito e all'azione politica e istituzionale un contributo rilevante, come bene ha messo in evidenza il Presidente del Senato nel Emiddio Novi - e non temo di poter essere smentito - è stato uno dei migliori figli di questo Paese e la sua scomparsa è stata una grave perdita, soprattutto per la sua Campania e la sua Napoli, luoghi in cui ha sempre vissuto e che ha amato al pari della sua Sant'Agata di Puglia. Emiddio Novi ci lascia un'eredità importante e preziosa: il senatore Novi ci lascia i frutti fecondi del suo lavoro, i suoi scritti e le sue profonde riflessioni, ma ci lascia soprattutto una testimonianza, quella della vita di un uomo, di un intellettuale che ha saputo indagare profondamente e proficuamente nelle complessità del nostro tempo che con il suo impegno per gli altri, per la sua famiglia, per i suoi concittadini e per il suo Paese ha saputo dare un senso davvero alto alla propria vita e non solo. Alla moglie, ai figli e a quanti, come noi, l'hanno conosciuto e frequentato va il senso più profondo della nostra vicinanza. A lui, al nostro amico Emiddio, va il nostro più profondo senso di gratitudine. Ciao, Emiddio.

Signor Presidente, oggi ricordiamo il senatore Emiddio Novi, che è stato in Senato a lungo che è scomparso nello scorso agosto in circostanze che tuttora tanti stentano ad accettare. Io l'ho conosciuto nel 2003, quando sono stato eletto per la prima volta in Senato, oggi lo commemoro con quel sentimento di colleganza che dovrebbe sempre legare tutti noi, a prescindere dai rapporti politici che possono vederci alleati o avversari. Emiddio Novi era un senatore politicamente molto impegnato, ma anche riservato e silenzioso, ed è per questo suo tratto che ci siamo conosciuti solo da lontano, guardandoci, lui seduto nella parte destra dell'emiciclo e io nella sinistra. In tanti anni non ricordo di avere mai avuto con lui una conversazione personale. E lo dico con rimpianto, per un modo di stare in una stessa Aula, che talvolta ci riguarda e ci vede passare giornate nello stesso luogo senza mai rivolgerci personalmente la parola. Ed è uno dei tanti dati che rendono difficile questo nostro tempo e ci fanno temere le conseguenze di tanta incomunicabilità. Sia pure da lontano, però, l'ho osservato e seguito, apprezzando, non soltanto il suo impegno a favore di una moratoria universale delle esecuzioni capitali, ma anche l'assiduità con cui frequentava l'Aula del Senato e l'impegno politico coerente nei confronti delle posizioni del suo Gruppo. Commemorare Emiddio Novi mi permette di dire che un modo alto di ricordarlo dovrebbe essere quello di impegnarci, tutti noi senatori, ad un autentico rispetto reciproco, cercando sempre di non trasformare il dissenso politico in una inimicizia e di non considerare l'avversario politico un nemico da abbattere con ogni mezzo, consentito o non che sia. Gli eccessi d'Aula e le volgarità alle a tutti noi è capitato di assistere sono un segno di decadenza e di malcostume che fanno ben poco onore alla dignità del Parlamento. Il Parlamento italiano nelle ultime legislature ha perso molto del prestigio e dell'autorevolezza che ha avuto nei decenni. Questo non fa bene alla democrazia. Dobbiamo recuperare la civiltà del confronto tra di noi, facendo valere i nostri argomenti e non cercando di imporre le nostre intemperanze, dobbiamo ricordarci che la politica si fa con la testa e non con la pancia. Permettetemi un accenno a qualcosa di grande di cui abbiamo avuto notizia negli ultimi giorni e che, in fondo, riguarda anche noi. Nei giorni scorsi ho seguito le commemorazioni con le quali negli Stati Uniti è stata onorata la scomparsa del senatore repubblicano JohnMcCain. I discorsi in ricordo di McCain che più mi hanno colpito sono stati quelli di due democratici, due suoi avversari politici, il senatore Joe Biden, ex Vice Presidente, e l'ex presidente Barack Obama. Negli interventi di Barack Obama e Joe Biden spiccavano il rispetto, l'ammirazione e la considerazione con cui ricordavano quello che era stato un *leader* e un loro fiero ma leale avversario politico. Obama e Biden mi hanno più volte fatto pensare a noi, alla nostra incapacità di onorare e rispettare i nostri avversari politici, di riconoscere i meriti e anche, quando ce l'hanno, le ragioni. Nel ricordare oggi il senatore Emiddio Novi, anche memore di un avversario con il quale mai ci sono stati scontri politici non ortodossi, voglio pensare che il Senato torni ad essere un luogo di confronto sempre civile delle idee e delle piattaforme politiche e che mai ceda alle tentazioni di risolvere i problemi con l'insulto e con le offese reciproche.

Signor Presidente, grazie per avere voluto ricordare oggi qui Emiddio Novi. Egli è stato un collega appassionato, generoso e coerente; un uomo che non si è mai nascosto nelle sue battaglie politiche, che le ha sempre fatte a viso aperto, che ha saputo anche essere divisivo nel suo impegno politico. Ma tutto questo non è mai venuto meno rispetto alla sua capacità di essere leale con gli altri. Chi mi ha preceduto ha ricordato la nobiltà della politica, quella che dovrebbe essere nobiltà. Fa parte di un rito, ricordare una persona che se ne è andata e che è stata seduta in quest'Aula? Io credo di no: fa parte di un momento alto di quest'Assemblea e della politica, perché una democrazia vive e si arricchisce anche con la memoria di chi è passato da qui, con la memoria di chi ha dato il suo contributo. Io l'ho avuto come collega, ne ho apprezzato la capacità politica, la cultura e la profonda umanità. Per lui non ci sono stati degli avversari come nemici, ma degli interlocutori politici con cui aveva il gusto di coltivare anche un dialogo fuori dalla ufficialità di quest'Assemblea. Ecco perché, in questo momento, ricordo un galantuomo e con questa parola penso di riassumere le grandi qualità di Emiddio Novi ed è giusto che nelle forme e nei modi che si riterranno opportuni, d'accordo con la sua famiglia, a cui esprimo una condivisione profonda dei sentimenti di vuoto che egli ci ha lasciato, noi dovremmo trovare il modo di ricordarne la figura e il lavoro politico. *(Applausi).*

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi giovedì 6 settembre, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 4 ottobre. Il calendario di questa settimana prevede la discussione del disegno di legge istitutivo della Commissione di inchiesta parlamentare sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», nonché, ove concluse dalle Commissioni, delle proposte di inchiesta parlamentari monocamerali sul terremoto di L'Aquila e sul femminicidio. Domani, alle ore 9,30, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà un'informativa sulla vicenda della nave Diciotti. I Gruppi potranno intervenire per dieci minuti. Nella settimana dal 18 al 20 settembre sarà discusso in terza lettura, ove modificato dalla Camera dei deputati, il decreto-legge proroga termini, in scadenza il prossimo 23 settembre. Il calendario della settimana dal 25 al 27 settembre prevede la discussione, dalla sede redigente, del disegno di legge sull'obbligo di installazione di dispositivi di sicurezza per bambini nei veicoli, già approvato dalla Camera dei deputati, nonché i disegni di legge di rendiconto 2017 e assestamento 2018. Ove non conclusi, i predetti argomenti saranno esaminati nella settimana dal 2 al 4 ottobre. Il calendario dei lavori prevede inoltre, per ciascuna settimana, sedute di sindacato ispettivo e, ogni giovedì alle ore 15, il *question time*. Infine, il calendario potrà essere integrato con la discussione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, nonché con una informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale in relazione agli sviluppi della situazione in Libia. Su quest'ultimo punto la Conferenza dei Capigruppo si riunirà giovedì 13 settembre alle ore 9,30. Informo che la Conferenza dei Capigruppo ha preso atto delle nuove direttive disposte dalla Presidenza circa i criteri di redazione degli atti

le interrogazioni contenenti elementi estranei rispetto alla «semplice domanda rivolta al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare

Entrambe le disposizioni appaiono inequivoche nel collegare la funzione degli atti di sindacato ispettivo alla concreta sfera di competenza dell'Esecutivo. Pertanto, interrogazioni e interpellanze volte a chiedere l'intervento del Governo in ambiti ad esso preclusi (come le competenze guarentigiate di organi costituzionali, attribuzioni di altri poteri dello Stato, autorità indipendenti, ovvero organi territoriali o sovranazionali, attività di partiti politici) saranno considerati improponibili ai sensi delle predette disposizioni regolamentari. Alla luce dei predetti criteri, la Presidenza ritiene opportuno fissare un limite anche in termini dimensionali alla redazione degli atti di sindacato ispettivo che dovranno essere contenuti al massimo in due cartelle.

Signor Presidente, colleghe e colleghi senatori, il disegno di legge n. 536 d'iniziativa della senatrice Bottici e di altri, che oggi siamo in quest'Aula chiamati a votare, prevede la costituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto». La proposta in esame riprende il contenuto dell'atto del Senato 2030 approvato nella scorsa legislatura in prima lettura dal Senato. Il testo, approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia, è stato modificato nel corso dell'esame in sede redigente, con l'approvazione di tre puntuali emendamenti presentati dalla sottoscritta relatrice. Prima di procedere alla disamina del provvedimento, è opportuno dare conto, seppure sinteticamente, dei fatti gravissimi sottesi alla proposta di costituzione di una Commissione di inchiesta. La cooperativa agricola «Il Forteto», comunità di recupero per minori disagiati sita nel Comune di Barberino di Mugello, in Provincia di Firenze, è stata al centro di una lunga vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti e pedofilia, iniziata già alla fine degli anni Settanta, culminata nel 1985 con una prima condanna definitiva dei cofondatori per maltrattamenti aggravati e atti di libidine. Si tratta di Rodolfo Fiesoli, detto il «profeta», e di Luigi Goffredi. Vicenda conclusasi nel 2015, per Fiesoli, con un'ulteriore condanna (in primo grado) a diciassette anni di reclusione, ridotta a quindici anni e dieci mesi in appello, per violenza sessuale e maltrattamenti. Quest'ultima sentenza è stata impugnata in Cassazione. La suprema Corte nel 2017, con la sentenza n. 3346, ha reso definitiva la condanna di Fiesoli, annullando con rinvio limitatamente ad uno degli episodi di violenza sessuale. Per gli altri nove imputati, compreso Goffredi, pur avendo dichiarato i reati estinti per prescrizione, ha confermato le relative statuizioni civili. Successivamente alla sentenza del 2017, la vicenda giudiziaria ha avuto ulteriori sviluppi (non richiamati nella relazione illustrativa). In relazione all'ordine di esecuzione della pena, emesso nel il Fiesoli ha proposto richiesta di annullamento alla corte d'appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione per impossibilità ad eseguire una pena che non ha i caratteri di certezza e irrevocabilità. La corte fiorentina, nel gennaio 2018, ha rigettato questa richiesta con ordinanza. Infine tale decisione, impugnata in Cassazione, è stata annullata senza rinvio dalla Suprema corte (sentenza n. 30780 del 2018), con conseguente provvedimento di revoca dell'ordine di esecuzione che era stato emesso dalla procura il 23 Ebbene, ancora oggi Fiesoli si trova in stato di libertà, con conseguente rabbia e sgomento di tutte le vittime e dei loro familiari. Sennonché, seppure già nel 1997 Fiesoli avesse una condanna gravissimi capi di imputazione, risultava ancora a capo della comunità e - come si precisa nella relazione di accompagnamento del disegno di legge - il tribunale dei minorenni continuava ad affidare minori alla struttura: si contano 60 minori affidati alla struttura fino al 1990. Proprio per il trattamento subito dai due bambini affidati dal tribunale dei minorenni alla comunità «Il Forteto» - intanto divenuta anche cooperativa agricola con l'acquisizione di 500 ettari nel Comune di Dicomano, sempre in provincia di Firenze - l'Italia è stata condannata nel luglio del 2000 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza Scozzari e Giunta contro Italia n. 39221 del 2000), adita dalle madri alle quali i minori erano stati tolti. è stata condannata a pagare una multa di 150 milioni di lire come risarcimento dei danni morali. Più nel dettaglio, nel settembre 1997 due bambini nati nel 1987 e nel 1994, di cui le ricorrenti erano rispettivamente la madre e la nonna, venivano inseriti con provvedimento giudiziario nella comunità «Il Forteto». Si legge nella sentenza: «Due dei principali dirigenti e fondatori della comunità erano stati condannati per aver abusato sessualmente di tre handicappati affidati alla loro custodia, fatti noti ai giudici interni. Prima dell'inserimento in comunità, il maggiore dei due bambini era stato vittima di violenza di natura pedofila da parte di un operatore sociale». La corte ha giudicato che i due dirigenti incriminati incriminati avevano svolto un «ruolo attivissimo» nella custodia dei minori e ha concluso che vi era stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (per la precisione, del diritto al rispetto della vita privata e familiare) a causa, in particolare, dell'affidamento ininterrotto di questi alla comunità «Il Forteto».

nell'agosto 2013 ne ha chiesto il commissariamento (richiesta successivamente respinta dall'assemblea della cooperativa), motivandolo a causa della pesante e invasiva commistione tra la comunità e la cooperativa agricola direttamente coinvolta nella gestione degli affidamenti dei minori e disadattati. È proprio dell'altro giorno la dichiarazione delle sigle sindacali FLAI CGIL, che si dicono fortemente preoccupate della commistione tra l'azienda e la comunità. Ebbene, il disegno il disegno di legge che ci apprestiamo a votare consta di 9 articoli. L'articolo 1 prevede, così come modificato dalla Commissione, che sia istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta bicamerale sui predetti fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», con il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti di minori, al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura. I compiti della Commissione, enunciati nell'articolo 1, sono poi puntualmente indicati nell'articolo 2, anch'esso modificato dalla Commissione. Si legge che la Commissione è chiamata ad accertare i fatti e le ragioni «per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiamo proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunità «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte» perpetrate all'interno della comunità; nonché a verificare i «presupposti per la nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura «Il Forteto» inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento». Il disegno di legge attribuisce, poi, alla Commissione il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale, al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo a essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori. La Commissione, ai sensi dell'articolo 3, sarà composta da venti senatori e venti deputati, nominati dai rispettivi Presidenti, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo. Compete alla Commissione stessa l'elezione dell'Ufficio di Presidenza (Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari). Il comma 2 prevede che i componenti della Commissione dichiarino alla Presidenza della Camera di appartenenza di non aver ricoperto ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta. Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, l'articolo 4 prevede l'adozione da parte della Commissione di un regolamento interno. Relativamente ai poteri, l'articolo 5, comma 1, prevede che la Commissione proceda all'espletamento dei suoi compiti con gli stessi poteri di indagine e istruttori e con le stesse limitazioni Per i segreti di Stato, di ufficio, professionale e bancario, ai sensi del comma 2 trovano applicazione le norme vigenti e la legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché l'articolo 203 del codice di procedura penale. Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, l'articolo 5 dispone l'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 366, relativo al rifiuto di di uffici legalmente dovuti, e 372 del codice penale, che punisce la falsa testimonianza (articoli di cui al Capo I, Titolo III del Libro II del codice penale). Il comma 3 dell'articolo 5 disciplina la richiesta di atti e documenti, prevedendo che la Commissione possa richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, anche se coperti da segreto, procedendo contestualmente al mantenimento del regime di segretezza per tutti gli atti e i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari custoditi, prodotti, o comunque acquisiti da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione in materia attinente alle finalità dell'inchiesta. In tali casi, l'autorità giudiziaria deve provvedere tempestivamente, potendo ritardare la trasmissione degli atti richiesti solo per ragioni di natura istruttoria e con decreto motivato (decreto che ha efficacia per sei mesi ed è rinnovabile). La Commissione, inoltre, può ottenere da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da questi custoditi, prodotti o acquisiti in materia attinente alle finalità dell'inchiesta (articolo 5, comma 5) e richiedere copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia (comma 8). La Commissione può poi stabilire, in base al comma 6, quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti a istruttorie o altre inchieste in corso, mentre si prevede che debbano in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Il comma 7 precisa poi che è sempre opponibile il segreto tra il difensore e la parte processuale nell'ambito del mandato. Il comma 4 statuisce che il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione di inchiesta può essere opposto all'autorità giudiziaria.

L'articolo 6 del provvedimento disciplina l'obbligo del segreto per tutto ciò che attiene agli atti e ai documenti per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione e ogni altra persona che collabori con essa, compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. La violazione di questo obbligo è sanzionata penalmente ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. L'articolo 7 prevede, inoltre, che le sedute della Commissione siano pubbliche, salvo che la Commissione non ritenga opportuno deliberare di riunirsi in seduta segreta. Per il funzionamento della Commissione è fissato un limite di spesa pari a 50.000 euro annui; tali spese sono poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali. L'articolo 8, emendato sempre dalla Commissione, stabilisce che la Commissione di inchiesta deve completare i lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione e presentare alle Camere, nei trenta giorni successivi alla fine dei lavori, la relazione conclusiva della sua attività di indagine. L'articolo 9, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Ho concluso. Ringrazio il Presidente e l'Assemblea tutta.

Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, Rodolfo Fiesoli, il fondatore della comunità per minori maltrattati «Il Forteto» di Vicchio, in provincia di Firenze, al centro di varie inchieste per maltrattamenti e violenza sessuale, è stato scarcerato a seguito di una decisione della Cassazione del 5 luglio scorso. Fiesoli e il suo braccio destro Luigi Goffredi (per lui condanna a sei anni annullata per prescrizione) erano già stati arrestati nel 1978, pochi anni dopo la fondazione della comunità, per atti di libidine violenti e maltrattamenti su minori disabili e definitivamente condannati nel 1985. Eppure la voce delle vittime è rimasta inascoltata fino al 2011, quando Fiesoli è stato di nuovo arrestato e la procura di Firenze ha ripreso, con enorme fatica e tra pesanti diffidenze, a scavare negli orrori della comunità. nessuno poteva dire di ignorare le mostruosità del Forteto, eppure Fiesoli e Goffredi per decenni hanno gestito la comunità dove i minori venivano plagiati, sfruttati e abusati; «un'esperienza drammatica, a tratti criminale», dicono le carte processuali. Ma la sentenza coinvolge un intero sistema di potere in Toscana, fatto di complicità sottaciute e appoggi espliciti, di «corto circuito istituzionale», «strumentalizzazione» e una «linea di credito illimitata» aperta da Regione, Comuni rossi del Mugello, tribunale per i minorenni, servizi sociali, galassia coop. «Il Forteto» è una comunità di accoglienza ma anche una coop agricola rossa, tuttora funzionante, dove i minori accolti erano mandati a lavorare. Ha ottenuto finanziamenti e crediti, i suoi capi erano invitati a convegni importanti per spiegare il modello «educativo», la giustizia minorile continuava a inviare sul Mugello bimbi tolti alle famiglie che precipitavano in un abisso di violenze morali, fisiche e sessuali. Ma chi comandava in Toscana parlò di complotto ed errore giudiziario. Tribunali, servizi sociali, i partiti che governavano e foraggiavano generosamente «Il Forteto» con denaro pubblico (molti vip del partito chiudevano sul Mugello le loro campagne elettorali) hanno fatto credere che Fiesoli e compagni fossero i portatori di un'eccellenza educativa; ma il loro metodo era denigrare i genitori naturali, insegnare che il rapporto tra uomo e donna è impuro, fare il lavaggio del cervello ai piccoli ospiti. I ragazzi presi in affido venivano assegnati non a una coppia vera, ma a due genitori funzionali intercambiabili. L'omosessualità era presentata come liberatrice dalla materialità. Il «profeta», come veniva appellato Fiesoli, aveva rapporti sessuali con bambini e adulti; «Il Forteto» era il suo territorio di caccia, come hanno scritto i giudici. Nonostante questi fatti, finalmente acclarati, e una condanna a quindici anni e dieci mesi di reclusione, Fiesoli è tornato libero. Le reazioni delle vittime, dell'opinione pubblica e soprattutto del Parlamento non possono farsi attendere, perché questa scarcerazione è una vergogna. Il conformismo culturale e amministrativo è stato determinante affinché le violenze e gli abusi a «Il Forteto» si protraessero per oltre trent'anni, e bisogna agire affinché fatti simili non accadano mai più. Oggi, in quest'Assemblea, chiedere l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, sulla comunità «Il Forteto» significa accertare le motivazioni per cui le autorità giudiziarie interessate - comprese quelle investite di poteri di vigilanza - e le pubbliche amministrazioni, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale questa comunità, anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte all'interno della comunità stessa.

soprattutto per sottolineare a quest'Assemblea che il secondo comma dell'articolo 2 è un po' il cuore, a nostro avviso, dell'attività che deve essere svolta dalla istituenda Commissione.

sia per l'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale sia per il potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affido

tra Barbiana e Rossoio c'è una differenza abissale. C'è solo un punto in comune e lo sottolineo, perché ho letto che il signor Fiesoli si paragonava a Don Lorenzo Milani. L'unico punto in comune è la distanza geografica: Barbiana dista da Rossoio pochissimi chilometri, forse nove. Il Comune di Dicomano non è Barberino di Mugello; anzi, una parte della tenuta è a cavallo fra i Comuni di Vicchio e di Dicomano: questo è l'unico punto sul quale possiamo significare una relazione tra questi due nomi. Definirei blasfemia - e lo dico da laico - l'accostare Don Lorenzo Milani accanto alla storia di Fiesoli e degli accoliti di quella che le carte dimostrano essere stata in perfezione una setta. Quelle sono anche le terre di Giotto: Giotto aveva lì una parte delle sue proprietà, ma nulla di ciò che la storia ha raccontato di recente fa sì che possano essere collegate a quella storia artistica. L'unico che può essere citato magari è il genio folle di Bosch quando parliamo della Dobbiamo avere la forza di chiedere non solo scusa alle vittime, che ancora oggi sono vittime di una storia tragica; spero che la formazione della Commissione di inchiesta, che la senatrice Bottici ha promosso ormai da molto tempo, sia anche l'occasione, non dico per mettere la parola fine alla verità, ma perlomeno per ricostruirne delle parti, che peraltro sono già state affrontate dalle e invito i colleghi senatori a leggerle, perché è una lettura significativa - che sono state rilasciate dalla commissione di inchiesta del Consiglio regionale della Toscana, qui citate dalla nostra relatrice. I fatti sono di una complessità e di una semplicità esemplare. Si tratta di una sorta di terrificante esemplare. Si tratta di una sorta di terrificante groviglio nel quale nessuna delle istituzioni può essere considerata o può considerarsi marginale:

sto parlando di apparati dello Stato che avrebbero dovuto vigilare e controllare, mentre direi che non lo hanno assolutamente fatto. Non c'è un dato che emerga dall'inchiesta della Regione che possa essere annoverato nel luogo della certezza e della verità: non il lavoro fatto per controllare chi vi lavorava. Siamo di fronte ad uno sfruttamento vero e proprio di chi lavora all'interno di quella cooperativa; siamo di fronte al lavoro nero, al lavoro senza nessun tipo di versamento legato a regime pensionistico e così via. Il termine da usare è «sfruttamento», senza nessun altro tipo di aggettivo. Vi sono poi i conflitti che si sono progressivamente manifestati e sono venuti alla luce tra i diversi livelli giudiziari:

è spingere affinché non possa essere escluso, con la rapidità che i tempi della tragedia richiedono, un commissariamento di quella struttura.

ancora oggi in quella cooperativa lavorano fianco a fianco le vittime e chi ha abusato di quelle donne e di quegli uomini. Parlare di commissariamento significa quindi fare una cosa santa e giusta. Dunque, fra le altre attività della Commissione, io suggerirei anche quella di lavorare perché questo obiettivo possa essere raggiunto quanto prima.

siamo oggi a discutere qui di una vicenda per la quale, se non fosse per la serietà della sede istituzionale in cui siamo, qualcuno potrebbe considerarci dei pazzi. «Il Forteto» è una di quelle storie vere che, se la racconti per strada, al bar o in altri luoghi ordinari frequentati quotidianamente, le persone stentano a credere che sia realmente accaduta. Dunque, cerchiamo di fare un po' d'ordine: c'è un luogo dove per trent'anni sono stati accolti minori in affidamento da famiglie con gravi problemi, dove sono stati commessi gravi abusi sessuali e violenze su minori. Un luogo dove maschi e femmine dormivano in aree separate in nome di una purezza dei rapporti intimi che induceva di fatto all'omosessualità, voluta e predicata da Fiesoli, il pedofilo capo di questa comunità. Ma soprattutto è stata una setta totalizzante in cui si è annullata la personalità dei soggetti, di ragazzi con gravi problemi, e si sono rovinate decine, centinaia di famiglie e di persone, perché a «Il Forteto» non ci sono stati soltanto gravissimi abusi su minori, le violenze, le botte e i rapporti sessuali completi messi in atto da Fiesoli. In quel luogo bambini che venivano fatti alzare all'alba per andare a lavorare, prima di essere portati a scuola, per fare un formaggio che magari mangiavano gli ospiti illustri - tanti, da politici a magistrati - che hanno frequentato la struttura. Da quel luogo non si poteva uscire liberamente. Chi ci lavorava non percepiva uno stipendio ma poteva disporre solo di una cifra minima. Tutto il resto rimaneva in cooperativa. Tutti i contatti con l'esterno venivano annullati in un sistema che plasmava la personalità e creava una realtà parallela che ha reso un inferno l'inserimento delle persone che ce l'hanno fatta (perché c'è anche chi non ce l'ha fatta ad uscire da quel luogo). In questo luogo è stato permesso di tutto nel silenzio e con la connivenza della politica, della magistratura, dei vertici socio-sanitari, con l'avvallo e l'aiuto della Regione Toscana che per anni ha considerato «Il Forteto» un esempio, finanziandolo e promuovendolo: tutto provato da sentenze definitive e dalle relazioni delle due commissioni regionali di inchiesta istituite dal Consiglio regionale della Toscana. Fiesoli, alla fine degli anni Settanta, finì in carcere per aver molestato sessualmente un disabile in presenza di un minore. la magistratura e le istituzioni conoscevano questi fatti che avrebbero dovuto suggerire quantomeno un principio di precauzione nei confronti di quest'uomo, se così lo vogliamo chiamare. Invece hanno deciso scientemente di ignorarli. Così, con l'avvio delle indagini e il nuovo arresto del dicembre 2011, Fiesoli, dopo sei anni di *iter* giudiziario, è stato nuovamente condannato in via definitiva il 22 dicembre 2017 dalla Cassazione per maltrattamenti e abusi sui minori. Nonostante questi fatti siano provati, oggi non è in carcere, perché ancora non si conosce l'entità esatta della pena. Per uno dei capi d'accusa, infatti, si deve ripetere il processo. Ma è possibile, mi chiedo e ci chiediamo, che per un pedofilo condannato per reati così gravi, il nostro sistema non preveda la galera senza se e senza ma? Mentre non c'è appello per le centinaia di vittime della comunità «Il Forteto» che hanno subito di tutto? E poi, stando alla giustizia, pare che in questa setta nessuno abbia collaborato con Fiesoli, nessuno, in trent'anni, abbia visto o abbia saputo cosa stesse succedendo. Delle 23 persone rinviate a giudizio in primo grado, nessuno è stato condannato in terzo grado: tutti salvi, perlopiù grazie alle prescrizioni sopraggiunte; persino quello che è stato considerato il braccio destro, l'ideologo Luigi Goffredi, condannato a otto anni in primo grado e a sei in appello, l'ha fatta franca. Questo quadro, cari colleghi, ci dice in maniera chiara ed inequivocabile che l'*iter* giudiziario non basta a mettere la parola fine su questa vicenda, intanto perché questo luogo esiste ancora ed è sempre lì, a Vicchio, nel Mugello. Molti dei processati e dei prescritti ci vivono e lavorano tutt'oggi, magari accanto alle persone che hanno avuto il coraggio di denunciare, e fanno il bello e il cattivo tempo. La cooperativa agricola ha tentato di mostrarsi una cosa diversa dalla comunità. Le stesse sentenze hanno messo nero su bianco, in modo inequivocabile, il fatto che cooperativa e comunità, negli anni, sono stati, invece, la stessa cosa, di amministrazione ci sono personaggi che hanno testimoniato in difesa di Fiesoli nei vari procedimenti giudiziari. Dunque, dobbiamo chiederci come è possibile che sia successo tutto ciò. Chi ha protetto Fiesoli? È possibile che i magistrati, i politici e gli operatori che hanno avuto a che fare con «Il Forteto» abbiano agito tutti in buona fede? È possibile che nessuno si sia accorto di nulla? Oggi, grazie all'ottimo lavoro dei magistrati di Firenze che hanno messo alla sbarra i responsabili dopo le fondamentali quanto coraggiose denunce delle vittime, sappiamo cosa è stato e cos'è «Il Forteto», ma non sappiamo abbastanza perché le stesse inchieste del Consiglio regionale della Toscana, approvate all'unanimità dopo un lavoro fondamentale in questa vicenda - è bene ricordarlo - si sono fermate di fronte a dei muri che sono sembrati insormontabili. Per questo, permettetemi di ringraziare tutte quelle donne e quegli uomini che hanno cercato di rompere questi muri. Un particolare ringraziamento lo voglio fare agli amici giornalisti Duccio Tronci e Francesco Pini per il loro libro inchiesta. Noi oggi dobbiamo provarci con una Commissione di inchiesta che ha il dovere morale di tentare ogni strada per far luce su questa terribile vicenda, dopo anni di muri della sinistra Toscana che ha cercato in ogni modo di minimizzare e silenziare l'eco di questa storia, fino ad oggi sin troppo taciuta. Perciò, consentitemelo, mi viene da chiedere: cosa hanno da nascondere? Cosa avevate da nascondere? Con la maggioranza che oggi si è formata e che è presente in questo Parlamento abbiamo l'occasione di dare verità alle vittime e di risarcirle moralmente, laddove materialmente purtroppo non è più possibile. Per tutto quanto esposto, annuncio convintamente il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

Care colleghe e cari colleghi, oggi votiamo l'istituzione di questa Commissione di inchiesta sui terribili, indegni e ignobili fatti accaduti a «Il Forteto». Subito voglio esprimere a nome di tutto il Gruppo del Partito Democratico l'intenzione chiara, netta e forte del nostro voto favorevole. La vicenda della comunità di recupero «Il Forteto» è da anni - e purtroppo ancora oggi, l'hanno detto anche dei colleghi prima di me - una ferita aperta estremamente dolorosa per tutto il Mugello, per il territorio fiorentino da cui provengo, insieme ad altri colleghi, per tutta la Toscana - prima di me sono intervenuti e ormai anche per tutto il Paese, visto che siamo al Senato della Repubblica a parlarne e a interessarci di questo tema così difficile, doloroso e complesso. Gli orribili crimini che la magistratura ha accertato ci hanno colpito nel profondo, hanno scosso le nostre coscienze, hanno segnato tutto un territorio in questi anni, ma soprattutto hanno devastato, distrutto e segnato per tutta la vita le vittime alle quali, ancora una volta, esprimiamo tutta la nostra vicinanza. Il nostro partito ha affrontato e affronterà questo tema con l'attenzione e il rispetto dovuti a tutti coloro che hanno la vita segnata da abusi e violenze. Allo stesso tempo, però, staremo bene attenti a porci lontani e a bloccare qualsiasi strumentalizzazione politica di una storia così dolorosa. Non ce lo possiamo permettere. Ce lo impongono la nostra coscienza e la nostra responsabilità. Anche se la vicenda non è del tutto conclusa, come anche il senatore La Pietra e altri colleghi prima di me hanno ricordato, la magistratura ha emesso condanne in via definitiva. Partiamo, quindi, con un punto fermo: ci sono dei colpevoli individuati e riconosciuti. Attendiamo gli sviluppi dei processi e lo facciamo, ancora una volta, accanto alle vittime e alle loro famiglie,

pur restando ferma e netta la nostra fiducia nei giudici e nelle autorità competenti, ci impone di essere vicini con sensibilità a tutti coloro che sono stati colpiti in questa vicenda e da questa vicenda. La Commissione di inchiesta, per la cui istituzione voteremo oggi pomeriggio, deve essere un luogo per fare chiarezza, dare riconoscimento istituzionale a una pagina buia e terribile per il nostro Paese e formulare delle soluzioni, affinché attraverso la vigilanza delle autorità competenti sia limitata al massimo la possibilità che fatti orribili come quelli accaduti a «Il Forteto» non accadano in altre strutture analoghe e - oserei dire di più - perché non avvengano più in nessun luogo e non si possano replicare nelle strutture del nostro Paese. Due principi fondamentali guideranno il Gruppo del Partito Democratico all'interno di questa Commissione Il primo sarà il rispetto per il dolore delle vittime, che mai e poi mai permetteremo venga utilizzato in modo strumentale. Lo ribadisco con forza: non ce lo possiamo permettere. Il secondo sarà la tutela dei lavoratori e delle produzioni della cooperativa, così importanti per l'economia del territorio. È fondamentale infatti che si separi la vicenda della comunità «Il Forteto» da tutto ciò che di buono produce invece la cooperativa: non ci devono essere sovrapposizioni in questo senso. Per noi, per il territorio di riferimento, è di primaria importanza garantire i posti di lavoro e tutelare i lavoratori, slegando tutto quello che di orribile e ignobile è accaduto nella comunità fatti per i quali, lo ribadisco, i colpevoli sono già stati individuati e processati - dallo sviluppo di un'azienda strategica per l'economia di tante famiglie e di un intero territorio, quello mugellano, ma non solo. Presidente, colleghi, tutti sappiamo che alla politica, quindi a ciascuno di noi, è richiesta una responsabilità superiore quando si trattano argomenti che investono con forza l'esperienza umana delle persone. Con l'istituzione della Commissione in oggetto siamo chiamati a questo: abbiamo l'occasione, che spero nessuno di noi vorrà perdere, di dimostrare che la politica, quella con la «P» maiuscola, la capacità di essere attenta e responsabile, compatta e senza divisioni, nell'interesse di quei cittadini che ci hanno eletti Votando il disegno di legge in esame e preparandoci al lavoro in Commissione, mi appello quindi alla responsabilità di tutti noi - di ciascuno di noi, colleghi - perché riusciamo a portare avanti i nostri valori, non venendo mai meno a due principi: l'attenzione e la determinazione. Ci sono entrambe richieste e oserei dire imposte, affinché, senza rischiare di cadere in alcuna strumentalizzazione, si riesca a fare chiarezza, ad individuare i problemi e ad ipotizzare soluzioni che aiutino le istituzioni e le famiglie dei nostri territori. Se ci sarà l'impegno da parte di tutti i Gruppi a lavorare in questa Commissione con tale spirito, combinando in maniera equilibrata la sensibilità attenta imposta dalla vicenda e la determinazione responsabile a lavorare nell'interesse delle famiglie coinvolte e di tutto il territorio, allora il nostro impegno sarà all'altezza del ruolo che ci è stato affidato da chi ci ha permesso di essere in quest'Aula. Signor Presidente, è con questo spirito e con queste motivazioni

regionale, il segretario del PD di Firenze e il segretario cittadino del Mugello hanno espresso opinioni diverse, dicendo di no al commissariamento della struttura!

come sia potuta succedere una cosa simile in Toscana. Poi, signor Presidente, alla fine le darò la risposta che mi sono dato leggendo gli atti. Non vengo

Il pubblico ministero nella requisitoria finale, quando dice che in Toscana per decenni,

Vorrei richiamare l'Assemblea all'importanza dell'argomento che stiamo trattando. Ho già specificato che questa non è un'aula di tribunale, quindi qui non ci sono colpevoli ma si esprimono delle idee.

legislatura, vedendo poi sfumare tutto alla Camera, forse appositamente rallentato. La relatrice ha esposto fatti che forse non tutti hanno ascoltato, perché c'era un po' di disattenzione, ma hanno fatto male. È un peccato perché quello che è successo nella comunità «Il Forteto», nella sua atrocità, è purtroppo ancora adesso conosciuto da troppe poche persone.

A questo si è aggiunto un collasso delle istituzioni, una scomparsa dello Stato, una omertà che ha consentito il verificarsi di tutto quello che oggi è stato accertato da una sentenza di primo grado del tribunale di Firenze. In genere, nel dibattito politico e mediatico siamo soliti denunciare l'assenza dello Stato in relazione ad alcuni casi di criminalità organizzata, in alcune periferie in cui il potere delle cosiddette mafie (sappiamo cosa succede a Roma) è talmente forte che lo Stato, con le sue leggi e con i suoi poteri, sembra essersi ritirato. comunità «Il Forteto» però lo Stato, riferendomi in particolare alla cecità della magistratura e di alcune istituzioni, è completamente scomparso. In questo caso mafia e criminalità organizzata non c'entrano nulla e non c'erano guerre da combattere neanche sul piano militare; c'era una semplice comunità di persone organizzate in vari soggetti, tra cui una cooperativa agricola e una fondazione; una comunità all'apparenza pacifica, ma ai confini della quale sono state sospese per anni le leggi dello Stato. FI-BP)*. Sull'uscio di questa comunità ci si è fermati senza entrare, o forse senza approfondire, senza interrogarsi sul perché il «profeta» continuava a dirigere una comunità nonostante la prima condanna nel 1978 (Carlo Casini, magistrato in quel momento, iniziò a occuparsi del caso). Pertanto, né la politica, né le istituzioni, né i controlli dei servizi sociali si sono mai prese in prese in carico la responsabilità di accertare la verità che veniva denunciata dalle madri di alcuni bambini, e la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo lo dimostra. Insomma, all'interno di questa comunità c'era una zona franca da cui lo Stato aveva deciso di distogliere lo sguardo, di far finta che questa comunità, queste persone, ma soprattutto quanto avveniva in quel luogo, non esistessero. Già nel 1978, come è stato ricordato, Carlo Casini, che in quel momento non era ancora prestato alla politica, aveva aperto un'indagine esplicitamente rivolta a denunciare una serie di abusi che si verificavano nella Colleghi, stiamo parlando di quarant'anni fa e gli abusi che allora Carlo Casini denunciava erano esattamente quelli con cui oggi noi dobbiamo confrontarci. Non stupitevi del silenzio delle istituzioni, perché a quarant' anni da quello che è stato il percorso di inizio c'è ancora chi sostiene che lì non sia successo nulla di grave. In questi decenni, fino al 2010, si è continuato ad affidare minori e adulti in difficoltà a questa presunta comunità: 80 bambini e adolescenti, di cui 14 si sono suicidati e altri 8 sono morti tossicodipendenti, isolati, in uno stato di gravissima indigenza. Si è continuato senza che questa comunità ne avesse i requisiti e sapete perché? Perché non stiamo parlando di una casa famiglia, non stiamo parlando di una normale comunità. Questi bambini venivano affidati a pseudofamiglie, famiglie fittizie, finte, funzionali, come erano definite da questa comunità, che vietava rapporti eterosessuali, in cui donne e uomini dovevano vivere rigorosamente separati. Come è stato ricordato dal collega, nella sua requisitoria il pubblico ministero Galeotti, nel corso del processo ha detto: «In quella comunità si è verificata per anni una sospensione delle leggi dello Stato, tutto questo in un mare di omissioni, di silenzi, che oggi hanno contribuito a formare ombre gigantesche sulla vicenda da scacciare». E il tribunale dei minori di Firenze ha una gravissima colpa in tutto questo. Stiamo parlando di una comunità che è stata una sorta di Jekyll e Hyde, da una parte i premi, i riconoscimenti, i finanziamenti ricevuti dalla Regione Toscana per 1,254 le passerelle di importanti rappresentanti della sinistra italiana, D'Alema, Chiti, Camusso, Renzi. Ma nessuno se n'era accorto? Ad esempio nemmeno Pisapia, sindaco uscente di Milano, membro del collegio che patrocinò il «profeta» in Cassazione nel 1985 non ricordava e non ricorda Rosy Bindi, che più volte ha visitato «Il Forteto». Mi dispiace colleghi - e vorrei rassicurare la collega del Partito Democratico - ma non c'è strumentalizzazione politica in questa vicenda così atroce: noi vogliamo la verità e che ha commesso i fatti e chi ne era a conoscenza paghi il suo debito con la giustizia, come tutte le vittime, tutti i ragazzi hanno pagato per essere stati affidati a questo mostro. Tanti si dovrebbero vergognare. Mi ricordo anche quando, nella XVI legislatura, il Partito Democratico invitò Rodolfo Fiesoli in Senato a presentare il suo libro.

di controlli e di verifiche. Perché le denunce non venivano ascoltate? Dove erano gli assistenti sociali, gli psicologi, gli psichiatri, i controllori dei tribunali? E si continuavano ad affidare bambini. Nel 1985, dopo la prima condanna, Fiesoli esce dal carcere e nello stesso giorno viene affidato alla comunità un bambino affetto da sindrome di Down. Di questa vicenda stiamo parlando, colleghi, altro che di caccia alle streghe e strumentalizzazione politica. Entrare a gamba tesa: questo doveva essere fatto dallo Stato. Oggi questa Assemblea ha il dovere di assumersi la responsabilità, a nome di tutto il Paese, per le vittime di questi abusi, che sono stati comprovati, non inventati. È nostro dovere, prima per la nostra coscienza e poi per tutti coloro che rappresentiamo, e cioè gli italiani,

Questi ragazzi erano obbligati ad avere rapporti omosessuali come mezzo per la purificazione, dovevano rifiutare la famiglia di origine, la donna era considerata una meretrice che diventava schiava degli uomini per tutte le operazioni quotidiane. Erano obbligati ad avere rapporti con gli animali, avete capito bene? O Zoofilia, è tutto documentato. Nella comunità «Il Forteto» le aberrazioni avvenivano anche nei confronti dei disabili. Cito una testimonianza: «Ci mettevano di fronte a scene terribili, per farci vivere una sorta di terapia, secondo loro. Ricordo che una delle scene che mi ha spinto a uscire è stato vedere un ventottenne disabile psichico costretto a ingerire il mangime e le defecazioni delle mucche da una ciotola per cani. Vomitò e fu costretto a mangiare il suo vomito. I maltrattamenti servivano a terrorizzare le persone». Non è strumentalizzazione politica leggere le deposizioni dei testimoni. Andatevi a leggere le testimonianze. Altro che strumentalizzazione, sarei veramente sorpresa se in quest'Assemblea ci fosse qualcuno che non si senta in obbligo di votare a favore della istituzione della Commissione di inchiesta, perché credo che stia alla coscienza di tutti voler scacciare queste ombre. Questa vicenda non è una vergogna solo per «Il Forteto», non è una vergogna solo per la Toscana: è una vergogna per il nostro Paese e per questo ci chiama alla responsabilità. E mi auguro anche che la Commissione possa vigilare sulle condizioni dei lavoratori all'interno della casa famiglia, la cui normativa per ricevere permessi di apertura dovrebbe essere rivista *in toto*. Forza Italia voterà convintamente a favore dell'istituzione di questa Commissione (credo che nessuno avesse dubbi in proposito), perché deve essere fatta luce sulle tante ombre che sono state illuminate soltanto da una coraggiosa campagna di stampa

che, oltre ai colpevoli diretti, paghino il conto - e lo ripeto - tutti coloro che sapevano e che hanno taciuto. La speranza di tutti è che le persone che hanno tenuto questi comportamenti criminali e inaccettabili siano presto condannate definitivamente, senza cavilli giuridici, e che soprattutto

arriviamo qui oggi dopo anni di discussione. È vero che non dobbiamo utilizzare il dolore delle vittime per

pensando che sia stato normale che nessuno se ne sia accorto. Non è normale, perché quando il Fiesoli, nel 1979, viene arrestato

che sono cresciuti all'interno di questa cooperativa agricola. È una cooperativa agricola, non è una comunità è una comunità quella a cui venivano affidati i bambini; bambini che poi venivano subaffidati, all'interno dei soci, alle famiglie funzionali. E non si tratta del fatto dei rapporti omosessuali o meno. Erano costretti, è questo il problema, c'era una manipolazione della mente; è questo il fatto più terribile. Chi ha dato l'autorizzazione al Fiesoli, al «profeta», di fare un progetto educativo all'interno delle scuole (elementari, medie e superiori)? Chi sono i responsabili? Quali sono e dove sono? Hanno fatto carriera, non l'hanno fatta? Sono ancora all'interno delle istituzioni? Queste domande ce le dobbiamo porre. I minori che hanno seguito questo progetto educativo del «profeta» sono stati monitorati? Sappiamo se hanno subito danni? No, perché non ce lo possiamo chiedere. La Commissione di inchiesta parlamentare serve quindi a questo, perché nonostante

tutti coloro che sono entrati in contatto con loro - hanno subito un danno, perché un minore che subisce una violenza da adulto

a questo, ossia capire come mai i canali istituzionali non sono stati in grado di ascoltare e agire.

tratta di una realtà produttiva che anche oggi funziona. Noi dobbiamo separare quella che è stata la gestione

E allora c'è un motivo. Bisogna indagare sul perché e non sta a noi. Mi auguro che il Ministero inizi il percorso. So che sono già andati

potremo guardarci in modo migliore, perché siamo tutti colpevoli e responsabili. Opposizione e maggioranza devono oggi fare un passo in più e mettere

anni, se n'è andata la nostra collega della Camera dei deputati e nostra amica Iolanda Nanni. Iolanda ci ha lasciato in eredità, oltre al suo sorriso, un limpido esempio di attivismo civico, intraprendente e responsabile, ricco di sensibilità e passione. Prima di essere eletta al Consiglio regionale lombardo, nel 2013, era stata fondatrice e portavoce del Coordinamento provinciale pendolari della provincia di Pavia, la sua terra di origine, dove aveva portato avanti importanti battaglie su mobilità, ambiente, salute, beni comuni, pari opportunità. A settembre 2017, ad alcuni mesi dalla fine della X consiliatura in Regione Lombardia, che l'ha visita portavoce battagliera e determinata per quasi cinque anni, annunciava così il suo ritiro: «Mi scuso con tutti i cittadini pavesi e lombardi per non potermi più occupare di voi nei prossimi tempi. Ho gravi problemi di salute e devo combattere una battaglia personale contro un nemico infame, che da buona guerriera ho tutta l'intenzione di vincere e sconfiggere, per poi tornare, come sempre, al al vostro servizio». Riabilitatasi, aveva poi ripreso l'impegno politico con il Movimento ed era stata eletta a marzo scorso in Parlamento, contribuendo, con la sua solita tenacia, ai lavori della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati. Iolanda ci ha insegnato a non arrenderci, a cercare sempre la verità, a combattere al fianco dei cittadini. Ci lascia un'importante eredità: il suo esempio e il suo lavoro, da portare avanti con tutto il nostro impegno, per l'ambiente e per la salute di tutti.

Signor Presidente, intervengo a nome anche del mio collega, senatore Pittella, e di altri colleghi che hanno firmato l'interrogazione parlamentare Chiedo ai Ministri dei beni culturali, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione la risposta a un'interrogazione che assume, Presidente, carattere di urgenza perché riguarda 1.050 giovani che hanno svolto il servizio civile nazionale presso il Ministero dei beni culturali, che domani, 12 settembre 2018, terminano Queste ragazze e questi ragazzi, per avere accesso al bando, hanno dovuto superare una prova selettiva e in questo anno di durata del servizio civile hanno acquisito sul campo notevoli competenze, valorizzando anche il nostro patrimonio artistico, data la carenza di personale che c'è nel Ministero dei beni culturali, come ricordato anche dal Ministro. Il Ministro si è impegnato, alla Camera dei deputati, ad assumere personale. Questi nostri giovani meritano attenzione e di vedere riconosciuto e valorizzato il loro percorso, per farne tesoro in ambito formativo e lavorativo. Chiediamo urgentemente, quindi, ai Ministri, oltretutto nell'anno europeo del patrimonio culturale, come intendano valorizzare questo loro percorso, visto che la legge n. 106 del 2014 declina azioni concrete, e come non disperdere la pluralità di conoscenze e di competenze acquisite dalle ragazze e dai ragazzi nel corso dei progetti di servizio civile nazionale nazionale svolti all'interno del Ministero, visto anche che nella definizione dei bandi per le nuove assunzioni è prescritto per legge che è possibile prevedere come titolo di preferenza l'aver svolto il servizio civile universale. Presidente, rivolgo, tramite lei, un appello ai Ministri. La maggior parte di questi giovani volontari si è costituita in una rete e ha indirizzato una lettera al Governo. Il motto dell'Anno europeo del patrimonio è «Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro». Ecco, raccogliamo le speranze di questi ragazzi e rispondiamo al loro desiderio di futuro con azioni concrete.

su Genova e sulle necessità della città dopo la tragedia avvenuta. Genova è una città ferita; Genova non è un problema solo genovese o della Liguria, ma un tema nazionale, un'emergenza nazionale. Devo dire in questa Assemblea che trovo molto positivo lo spirito della città, che sta cercando di fare di tutto per rialzarsi con coraggio e abnegazione. e abnegazione. C'è un lavoro molto positivo fatto dagli enti locali in un'emergenza assoluta, come potete immaginare. Non parlo solo degli sfollati, ai quali si stanno trovando le case, fortunatamente, ma che vorrebbero recuperare almeno i loro oggetti più cari; non solo delle attività economiche: pensate a tutte quelle che si trovano nella zona rossa, completamente isolate e senza alcuna possibilità di avere le minime entrate che che permettano di andare avanti. Pensate al porto, alle attività industriali: la città è completamente separata e divisa.

le parti esistenti del ponte. Occorre creare rapidamente una viabilità alternativa sulla sponda destra e sinistra del Polcevera. Bisogna ripristinare le circolazione in corso Perrone; bisogna ripristinare la linea ferroviaria, che è centrale oggi. Il trasporto pubblico locale va potenziato, i servizi della sanità: oggi muoversi dalla Val Polcevera per chi, per esempio, ha un problema sanitario, con i tempi di percorrenza diventa drammatico, quindi vanno riorganizzate anche queste situazioni. Bisogna soprattutto ricostruire presto un nuovo ponte. Parlando un po' con tutti gli attori che stanno vivendo questa tragedia, quello che chiedono sono tempi certi, per per non perdere le attività economiche, per potersi risollevare. Quindi, penso sia importante non fare o vedere balletti ideologici, ma tutti insieme lavorare

con misure specifiche di carattere economico e fiscale e specifici ammortizzatori sociali per coloro che stanno perdendo il lavoro, per le imprese che non possono più dare lavoro a chi lavorava prima per loro. anche alla luce delle parole con cui abbiamo aperto questa seduta, ci sia la più ampia coesione di tutte le forze politiche per far sentire anche nei confronti del Governo la voce del Senato, che su questo chiede il massimo impegno e la massima rapidità.

Si tratta di una minore, che è stata messa per ben due volte in una sorta di casa famiglia, una volta in una comunità, poi in un'altra, e in entrambi i casi abbiamo sollevato il problema della risposta, della funzionalità di queste strutture ai bisogni reali dei minori e all'attenzione concreta dei loro genitori. Credo che se vogliamo dare valore al dibattito di oggi pomeriggio, non solo sulla gravità dei fatti accertati, ma sui silenzi pregressi che ci sono stati, occorre prendere maggiormente in

dei diritti dei minori e anche di eventi come quelli che abbiamo denunciato oggi pomeriggio, in modo così collegiale e nella piena condivisione di tutti,

Commissione di inchiesta sulla tutela dei minori. I minori non possono essere lasciati abbandonati all'indifferenza delle istituzioni, che sono uno strumento altrettanto drammatico della crudeltà, non solo di quel «profeta», ma di altre persone che

dovere, nell'immediatezza del crollo del ponte, di recarmi sul posto e interrompere tutto quello che stavo facendo (famiglia e vacanze). Lì ho visto una realtà che neanche in un film di fantascienza si può immaginare. Ho toccato però con mano la fierezza di essere a fianco a un Governo che ha fatto altrettanto: si è precipitato sul luogo dell'accaduto e ha detto immediatamente parole forti e coraggiosissime per

Noi, come tutti i parlamentari genovesi del MoVimento 5 Stelle, insieme ai Consigli regionali e comunali, abbiamo contribuito con proposte concrete, che siamo certi di vedere recepite in questo decreto-legge. Vigileremo in ogni caso affinché tutti gli enti - quindi Regione, Comune e anche il Governo - facciano tutto quello che deve essere fatto Il rischio è reale: Genova può recedere negli anni, perché oltre ai morti, oltre alla ferita simbolica, c'è un quotidiano logorio delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie. Quello che prima facevano in un certo tempo, lo fanno adesso con tempi raddoppiati, perché Genova è spaccata non in due, ma in quattro. La viabilità Nord-Sud ed Est-Ovest è completamente paralizzata. Quindi, ringrazio il Presidente che ha avuto parole di attenzione. Ringrazio il Governo e invito i parlamentari

la mia vicinanza a tutto il popolo genovese che è stato martoriato da questo evento tragico, che ha spezzato non solo una via di comunicazione, non solo le vite delle vittime,

Onorevoli colleghi, le Commissioni ambiente e affari costituzionali non hanno ancora concluso l'esame in sede redigente delle proposte di costituzione delle Commissioni parlamentari di inchiesta sul terremoto de L'Aquila e sul femminicidio,